L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

per il gesto di stizza che ho usato nel mio richiamo al Regolamento. A parte questo, vedo il Resoconto stenografico e non so se la censura è riportata anche nel processo verbale. Eventualmente le chiedo la cortesia di inserirlo.

rispetto a questo, chiedo che vada fatta chiarezza, perché il Presidente può assumere provvedimenti disciplinari, ma non può insultare nessuno dei senatori. Chiedo gentilmente di farsi da tramite con la Presidente del Senato affinché venga a chiedere scusa al senatore Santangelo e si eviti in futuro di rifare la stessa cosa. Non credo possano esserci dei provvedimenti disciplinari nei confronti del Presidente del Senato. Nella vita comune la Corte di cassazione ha sancito che si e lo ha condannato. Io mi auguro che anche il Senato lo consideri tale, e che, con la giusta onestà intellettuale che sicuramente il Presidente del Senato ha, possa venire a chiedere scusa, in modo da ristabilire un equilibrio sui fatti accaduti ieri.

all'articolo 5 e il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i relativi pareri. A questo punto dovremmo sospendere la seduta o, in alternativa, potremmo

apprezziamo le scuse che ha presentato alla Presidenza e all'Assemblea, ma abbiamo ascoltato gravi parole nei confronti della Presidente, che è stata accusata di aver insultato un collega. il senatore Santangelo ha richiesto provvedimenti disciplinari nei confronti della Presidente. Credo che ai più sia sfuggito, perché è accaduto nei primi minuti della della seduta e credo che i pochi senatori presenti non abbiano avuto modo di ascoltare. A fronte di questa richiesta - che noi riteniamo grave - di verifica ed esame del comportamento della Presidente, vorrei segnalare,

di quanto accaduto appena dopo la votazione sul cosiddetto disegno di legge Zan, che riprendeva i banchi del centrodestra. Quel video è stato inequivocabilmente fatto dai banchi del centrosinistra e credo che le posizioni fisse che abbiamo ripreso facciano facilmente individuare il senatore o la senatrice che ha fatto quel video. *(Applausi)*. Chiedo pertanto alla Presidenza

Grazie,

a un'aggravante rispetto alle pene detentive, per quanto concerne i funzionari pubblici. Ci appariva infatti sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione riferito alle responsabilità pubbliche, che già soggiacciono a precise sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di omissione o di colpa grave, per i quali l'interpretazione di questa norma potrebbe essere molto ampia, causando il proliferare di azioni penali ingiustificate nei confronti dei funzionari pubblici

le parole: «fermo restando il rispetto dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000»,

Signor Presidente, poiché tengo molto a questo emendamento 8.8, che mi invitano a ritirare,

a casa un'importantissima legge, la n. 132 del 2016, che istituiva nell'ISPRA e in tutte le agenzie territoriali un braccio armato ambientale per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente. La

Nell'intero bacino del Mediterraneo si sono registrati gravissimi incendi. Solo in Italia sono andati in fumo migliaia di ettari di territorio, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Calabria all'Abruzzo, dalla Campania alla Puglia e al Lazio; tutto con ingenti danni economici, minacce per l'incolumità delle persone e degli animali e ferite ambientali che si rimargineranno non prima di qualche decennio. Ogni attacco all'ambiente costituisce a tutti gli effetti un attacco alle fondamenta del nostro contratto sociale, soprattutto se, come dicono i numeri, la maggior parte degli incendi è di natura dolosa. Questi fenomeni criminali richiedono un consolidamento degli strumenti di prevenzione e controllo dei territori, nonché sanzioni più dure ed efficaci. Per questo, fra le tante misure introdotte, tengo a sottolineare le modifiche del codice penale, il costante aggiornamento dei piani regionali e il fatto che venga garantita alle strutture d'intervento un'adeguata capacità operativa. noi autonomisti è importante che questo nuovo impianto, con l'introduzione di nessi più stringenti tra il piano statale, quello regionale e il ruolo dei Comuni, si sviluppi senza intaccare le prerogative in materia di autonomie speciali, grazie alla clausola di salvaguardia approvata in Commissione.

Dispiace invece che la Commissione non abbia avuto la possibilità di apportare miglioramenti sostanziali dal punto di vista delle risorse economiche. In particolare, occorreva e occorre un intervento a favore dei territori più colpiti dagli incendi della scorsa estate, per la messa in campo di interventi di ripristino ambientale. Spero davvero che si trovino le risorse nella legge di bilancio, come richiesto da uno degli ordini del giorno approvati e com'è stato anche in qualche modo assicurato da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Per concludere, signor Presidente, oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento che ha soprattutto il merito di gettare le basi per evitare che la prossima estate sia come quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. Allo stesso tempo, accanto al miglioramento della *governance*, è necessario avere adeguate risorse economiche

con la legge di bilancio, ma anche con il PNRR, esattamente come indicato nel provvedimento, si rendano strutturali gli interventi per assicurare la sicurezza delle persone, dei territori, del patrimonio ambientale e degli animali. È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante l'estate di quest'anno i grandi incendi in Italia sono quasi triplicati rispetto all'anno precedente. un dato inquietante, che vuol dire in concreto che decine di migliaia di ettari di boschi e di macchia mediterranea sono andati distrutti, inceneriti dalle fiamme, alberi carbonizzati e oliveti e pascoli annientati. Tale situazione fa male all'ambiente, come pure all'economia. La spesa per far fronte agli incendi dell'estate scorsa ammonta addirittura a oltre un miliardo di euro i roghi creano gravi danni a flora, fauna, attività agricole, ambiente, biodiversità e spesso, purtroppo, anche agli insediamenti umani. Accanto a questi devastanti effetti immediati, ci sono poi pesantissime conseguenze a lungo termine, che compromettono l'intero ecosistema. Si tratta di danni per superare i quali bisogna investire mediamente almeno una quindicina d'anni, allo scopo di garantire il recupero delle aree, con costi estremamente ingenti. Per questo motivo è strategico investire in prevenzione, nel tentativo di intervenire in via anticipata, così da evitare gli incendi e i conseguenti disastri ambientali. Da qui, l'opportunità del provvedimento in esame, che ha il merito di prevedere misure aggiuntive immediate per la prevenzione, autorizzando il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno ad acquisire mezzi aerei e terrestri e strumentazioni utili a contrastare gli incendi boschivi già nell'anno in corso, attraverso un'azione mirata. prevede da subito lo stanziamento di fondi per il prossimo triennio, destinati agli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. risorse consentiranno di manutenere i boschi e le aree limitrofe, predisporre postazioni di atterraggio per i velivoli di soccorso e realizzare infrastrutture utili per gli interventi di spegnimento, come ad esempio le vasche di rifornimento idrico. Il provvedimento attribuisce inoltre alla protezione civile il compito di stilare ogni tre anni un Piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane e tecnologiche, creando così uno strumento utile a valutare in via anticipata criticità e soluzioni. Si tratta di un impianto normativo generale, che punta a rendere più efficace il contrasto. Gli incendi boschivi sono una piaga che mette a rischio il nostro patrimonio naturale, che si estende su un territorio molto vasto, se si pensa che più di un terzo della superficie italiana è coperta da boschi. Purtroppo, però, è un patrimonio fragile, che va tutelato, dal momento che è sempre più spesso vittima dei cambiamenti climatici, da un lato, e dell'azione dolosa dell'uomo, dall'altro. Ben sei incendi su dieci sono originati appositamente da piromani, come si è visto - purtroppo - nel corso dell'estate, quando sono stati numerosi quelli gravi appiccati in diverse Regioni del Sud (soprattutto in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia), provocando danni inestimabili. Significativo è il fatto che all'interno del provvedimento sia previsto anche l'inasprimento delle sanzioni, sia amministrative, sia penali, per i responsabili degli incendi dolosi. È giusto aver introdotto una nuova aggravante per i casi in cui ad appiccare il fuoco sia qualcuno che avrebbe avuto il compito di tutelare il territorio, così com'è positivo aver previsto che i dipendenti pubblici condannati per incendio doloso con una pena superiore ai due anni estinguano il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e siano interdetti dai servizi di lotta agli incendi. Insomma, si tratta di una legge con la quale lanciamo un messaggio chiaro all'opinione pubblica: chi provoca dolosamente un incendio commette un crimine e va punito di conseguenza. Non ci ha invece appassionato il dibattito, per tanti versi ideologico, che si è svolto in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali sul tema della possibile interruzione della caccia nei territori limitrofi a quelli nei quali è previsto lo stato d'emergenza a seguito di incendi gravi.

È cronaca di questi mesi, infatti, l'incremento massiccio di animali selvatici in diverse zone d'Italia, con una presenza che spesso mette a rischio il nostro comparto agricolo, nella misura in cui questi animali devastano le produzioni ortofrutticole dei nostri coltivatori e al contempo rappresentano - troppo spesso, purtroppo - una minaccia per la popolazione. Nell'anno dell'emergenza Covid, a causa dell'attraversamento di strade da parte di cinghiali o altri animali selvatici, si è verificato un incremento degli incidenti stradali (uno ogni due giorni), che hanno causato numerose vittime. Da qui l'esigenza di non introdurre norme che possano ulteriormente accrescere la presenza di animali predatori, come cinghiali, lupi o quant'altro. In sintesi, onorevoli colleghi, il provvedimento che votiamo oggi punta a ridisegnare la *governance* della prevenzione incendi e a potenziare la capacità operativa di coloro che sono impegnati nella lotta ai roghi. Questo provvedimento, purtroppo, non ha però a disposizione le risorse sufficienti per prevedere ristori per coloro che sono stati colpiti dalla forza devastatrice del fuoco. Per questo acquista ancora maggior peso l'impegno che il Governo ha assunto nei nostri confronti approvando un ordine del giorno di Italia Viva, fatto proprio anche dalle altre forze politiche, con cui si prevede che già nell'imminente legge di bilancio vengano stanziati aiuti specifici per le vittime degli incendi estivi, risorse che devono quindi servire innanzitutto ad assegnare i contributi a chi ha subito danni materiali dagli incendi. Serviranno poi a prevedere la sospensione del versamento dei tributi per chi vive nelle aree colpite, a rifinanziare il fondo regionale per la Protezione civile e a destinare ulteriori risorse a Regioni e Province autonome per l'acquisizione di nuovi mezzi operativi, sia terrestri che aerei. L'obiettivo è rendere possibile l'acquisto di strumenti innovativi satellitari, anche radar, videocamere, droni dotati di sensori, così da potenziare i sistemi di sorveglianza e di monitoraggio, perché l'innovazione al servizio dell'ambiente è la strada del futuro, se vogliamo tutelare il nostro patrimonio naturale; una strada che iniziamo ad intraprendere con questo decreto-legge. Nell'apprestarmi a concludere, signor Presidente, vorrei fare ancora un breve riferimento ad alcune considerazioni critiche che sono emerse durante la discussione generale in merito alla cosiddetta legge Madia dell'allora Governo Renzi. Pensare che gli incendi di quest'estate siano stati provocati dall'accorpamento del Corpo forestale sotto l'Arma dei carabinieri vuol dire prendere lucciole per lanterne e trattare i problemi del cambiamento climatico come se fossero un pranzo di gala. Certo che è sempre complesso razionalizzare e semplificare l'apparato pubblico, ma l'esperienza di numerosi altri Paesi europei dimostra che la lotta agli incendi è efficace ed è fattiva anche nella totale assenza di un Corpo forestale dello Stato. Stato. Signor Presidente, questo è il provvedimento meno opportuno per fare polemiche e strumentalizzazioni; serve invece compattezza delle forze politiche e del Paese per contrastare un fenomeno, quello degli incendi, di estrema gravità e complessità. e complessità. Noi vogliamo cogliere l'occasione del voto di oggi per esprimere in modo corale la nostra più sentita gratitudine a tutto il Dipartimento della protezione civile e al Corpo dei vigili del fuoco che, con grande spirito di abnegazione e senso dello Stato, si dedicano quotidianamente alla tutela del paesaggio messo in pericolo dagli incendi, senza risparmiarsi e senza esitare a mettere talvolta a rischio la loro stessa vita per il bene comune. Anche a loro oggi noi dedichiamo la votazione di questo provvedimento

la siccità, la desertificazione, i *record* negativi di pioggia che ci sono stati nei mesi scorsi erano delle avvisaglie di ciò che sarebbe potuto succedere. Non serviva sicuramente uno scienziato per capire che l'Italia sarebbe andata a fuoco, non a metà, ma tutta. Sono due i fattori che mancano e di cui il Governo non si è mai fatto carico: uno è sicuramente la prevenzione e l'altro è la manutenzione. alla prevenzione, avete smantellato i presidi sui territori e avete dimenticato soprattutto di coinvolgere i cittadini, che fanno una campagna attiva

al fatto che in Italia si bruciano i boschi soprattutto per creare discariche. Questo lo fa principalmente la mafia. Si bruciano discariche per creare altre discariche abusive. Ciò che fa rabbia e desta sconcerto è la sistematica

un decimo dell'energia che impegna per risolvere le lotte intestine avremmo, soprattutto in questa fase, una buona risoluzione dei problemi dei nostri concittadini.

che i terreni possano tornare ad essere di nuovo utilizzati. Per non parlare poi delle perdite, che non sono soltanto economiche, ma anche affettive della nostra comunità. Purtroppo la vastità del fenomeno ha manifestato, in maniera anche plateale, il fallimento. Ci sono stati infatti, signor Presidente, sicuramente dei fallimenti nell'organizzazione dell'Antincendio boschivo messo in campo sia dalla Protezione civile nazionale che da quella regionale. Il sistema degli appalti privati delle Regioni e anche soprattutto della Protezione civile governativa non solo è stato fallimentare, ma sappiamo che ha avuto anche È stato sicuramente un crimine depotenziare negli anni le flotte aeree dei Vigili del fuoco, della Polizia, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Forestale, dell'Esercito, della Marina e anche della stessa Aeronautica. Il vero problema è che non soltanto è stata

di un certo tipo di organizzazione e anche di alert preventivi adeguati. Ciò per noi sarebbe stato importante. Così come a più riprese abbiamo sottolineato la carenza dei Vigili del fuoco, dotati di pochissimi mezzi e, tra l'altro, con scarsa manutenzione. Perché abbiamo aspettato così tanto e perché devono verificarsi continuamente tragedie per assumere

soprattutto in questo periodo, se la manovra che in questi giorni sta impegnando il Governo e la maggioranza in una difficoltosa trattativa prenderà in considerazione questa drammatica situazione. Sentiamo parlare Sentiamo parlare di ulteriori stanziamenti per una misura che si è dimostrata fino ad oggi fallimentare ed anche puramente assistenziale, come il reddito di cittadinanza. Viene spontaneo chiedersi

Si antepone il reddito cittadinanza alla difesa dei boschi; sarebbe stato opportuno da parte del Governo pensarci prima, sicuramente non

guidato da Conte. Al tema delle risorse, che questo Governo continua, purtroppo, a non destinare, si aggiunge anche l'assurda soppressione - questa è la verità, Presidente - del corpo forestale dello Stato. Noi di Fratelli d'Italia diciamo da anni che è stata una scelta sbagliata; soprattutto, l'Italia è l'unica Nazione ad essersi privata del corpo forestale dello Stato, rinunciando così alla prevenzione e all'educazione ambientale, oltre che alla sicurezza. *(Applausi)*. Questo è sicuramente un momento particolarmente importante. Tutto ciò senza tener conto che l'implementazione delle politiche di prevenzione comporta anche una spesa decisamente minore rispetto a qualsiasi tipo di intervento in condizioni di emergenza.

i mali, la soluzione definitiva al problema: che sia solo un primo passo verso soluzioni di più ampia programmazione e anche di prevenzione. Ci auguriamo quindi che questo possa essere l'inizio di un percorso per arrivare a una soluzione. Per questi motivi, annuncio il voto di astensione del Gruppo

drammatiche che si sono ripetute quest'estate, che ci hanno mostrato i tanti disastri provocati dagli incendi. Incendi che hanno depauperato il Paese, il suo patrimonio naturale, il patrimonio boschivo e faunistico,

non solo per affrontare l'emergenza, ma per provare a mettere in campo un sistema di intervento e di prevenzione, che impedisca, già in un prossimo futuro, di dover constatare i danni che abbiamo dovuto contare in questa estate difficile. quindi di un provvedimento giusto e necessario, su cui - lo dico subito - il Partito Democratico voterà a favore.

chiarire bene e meglio quali devono essere le forme di coordinamento degli interventi di prevenzione e di lotta agli incendi. Occorre chiarire bene che il coordinamento deve avvenire tra tutti i soggetti interessati

la situazione che si verifica anno per anno. Allo stesso tempo penso sia molto importante che con il decreto-legge

gli strumenti di prevenzione e di lotta agli incendi, i mezzi e tutti gli strumenti tecnologicamente avanzati per poter anticipare il che gli incendi colpiscano ancora il Paese. Serve tutto questo, serve avere i mezzi e credo che il fatto che si stanzino 40 milioni di euro sia importante. Forse non è sufficiente, ma è un primo passaggio importante. Credo sia importante anche il fatto che, in sede di discussione della legge di approvato un emendamento presentato dalla presidente del Gruppo Misto, senatrice De Petris, che prevede l'utilizzo di droni e altre tecnologie per prevenire gli incendi e

dall'intervento umano e da interessi diversi, che convergono sull'idea di lucrare sugli incendi. questo è un altro tema importante di contrasto, insieme all'altro tema, sempre contenuto nel decreto-legge, che è quello delle sanzioni per chi provoca gli incendi e dell'aggravante per chi, pur dovendo stare dentro il sistema di prevenzione e lotta agli incendi,

francamente poco comprensibile su un tema che, con l'ordine del giorno votato prima,

c'è assolutamente alcuna volontà di contrastare i cacciatori o mettere in discussione la caccia. C'è un tema evidente, che riguarda la necessità di tutelare la fauna, anche di fronte a vicende così gravi come quelle degli incendi; si faccia senza penalizzare nessuno, ma assumendosi tutti la responsabilità di

per ridurre questo fenomeno drammatico, che depaupera quotidianamente il nostro Paese.

accogliere una serie di proposte che pure noi abbiamo avanzato; avremmo potuto rendere un servizio al nostro Paese cercando di dare un'impostazione diversa.

resta molto legato alla ricognizione dei mezzi, al monitoraggio. Penso, invece, che il salto di qualità che davvero dovremmo fare - e spero che si possa continuare a lavorare su questo - sia un vero e proprio piano, affidato a un'istituzione nazionale (va bene la Protezione civile), di prevenzione, di ricognizione, di lotta attiva, di strategia. Ci dobbiamo preparare al fatto che gli incendi boschivi, a causa dei cambiamenti climatici,

perché è una questione fondamentale. L'Italia è uno dei Paesi in Europa a più alto tasso di biodiversità e ha un patrimonio, dal punto di vista naturale, veramente importante. Se leggessimo

di prevenzione, ma serve anche accompagnarlo con un piano che sia davvero importante. Il piano forestale deve essere integrato e dobbiamo accelerare le misure

in una capacità non solo di coordinamento e ricognizione, ma anche di elaborazione di un vero e proprio piano strategico di prevenzione, lotta attiva e contemporaneamente di governo

il punto di innesco. Ovviamente è fondamentale anche per individuare i colpevoli, perché questo è l'altro problema: c'è una vera e propria industria del fuoco, è inutile che ci giriamo intorno. In questa industria del fuoco ci sono vari attori

È il motivo per cui, a mio avviso, oltre alla tecnologia - lo dico qui con chiarezza - non si è potuto fare un passo in avanti, per strane opposizioni.

tutti gli strumenti e le esperienze esistenti. Qui arriva un punto dolente: ho sentito prima una collega che diceva che qualcuno strumentalmente ha posto la questione del Corpo forestale. Ma quale strumentalmente? Quello è stato un errore, ce lo vogliamo dire o no? *(Applausi)*.

rappresentanti del Governo, colleghi, come hanno ricordato in molti, nel 2021 in Italia sono andati in fumo, avvolti dalle fiamme, 159.000 ettari di bosco, praticamente le città di Milano, Roma e Napoli messe insieme o di Venezia, Genova, Torino e L'Aquila. Abbiamo superato i 141.000 ettari del 2017, già *annus horribilis,* che, uniti ai 14.000 del 2018, ai 37.000 del 2019 e ai 53.000 del 2020, ci portano in vetta, un primato europeo in cui non vorremmo proprio più primeggiare. L'*escalation* di incendi della scorsa caldissima estate costa al Paese, secondo una stima di Coldiretti, circa un miliardo di euro tra opere di spegnimento, di bonifica, di ricostruzione. oggi la parola d'ordine non può essere che una sola: prevenzione. Investire sulla prevenzione significa risparmio in ogni senso: senso: innanzitutto di vite umane, di vite animali, di danni alle attività agricole e produttive, risparmio di risorse che potrebbero essere invece dedicate alla protezione del territorio e alla sua valorizzazione. Oggi dimostriamo in quest'Aula che questo Governo è riuscito a dare una risposta veloce al terribile fenomeno degli incendi boschivi, che ha funestato troppe Regioni italiane, soprattutto al Sud. Il decreto-legge contiene infatti misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro un fenomeno che rischia di degenerare e provocare danni irreparabili se non si attivano misure adeguate, efficaci e sinergiche tra gli enti di ogni livello, integrando e rafforzando il dispositivo normativo ed operativo esistente, come questo provvedimento si propone. Un piano di lotta agli incendi boschivi, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno diverse origini, dal comportamento inadeguato, quando non doloso, dell'uomo, alle condizioni meteo climatiche eccezionali. Intervenire durante e dopo un incendio divampato naturalmente significa dover assistere alla tragedia della distruzione di grandi parti di territorio, di vegetazione, di fauna selvatica, di animali domestici e da allevamento, di case, di attività, per non parlare delle vite umane. Riuscire a prevedere e a prevenire gli incendi significa evitare di arrivare tardi, significa tutelare - ribadisco - vite, attività e territorio. Oltre al piano di prevenzione, il decreto contiene anche disposizioni per sostenere e supportare le azioni per contenere gli incendi e limitare i danni che richiedono l'intervento di uomini, mezzi aerei e mezzi e mezzi terrestri, attraverso la predisposizione di strumenti ulteriori per favorire un coordinamento ancora più efficace tra i corpi dello Stato e gli enti del territorio. Proprio per questo mi fa piacere sottolineare come il Governo abbia saputo trovare quel punto di equilibrio tanto atteso tra competenze e responsabilità condivise tra Stato e Regioni, valorizzando la prospettiva inclusiva del sistema nazionale della Protezione civile e affidando al Dipartimento stesso della Protezione civile la funzione di coordinamento delle novità introdotte, per realizzare quella strategia di lungo respiro di cui tutti noi abbiamo parlato Sul fronte giudiziario, invece, viene messo a punto il dispositivo volto alla prevenzione e alla repressione dei reati di incendio boschivo e delle altre fattispecie commesse, perché i dati raccolti dai Carabinieri forestali testimoniano che solo il 2 per cento dei roghi ha una causa causa naturale, mentre il resto è provocato dall'uomo. Ben venga, allora, il rafforzamento del servizio nazionale della Protezione civile, ben venga il piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche aeree e terrestri necessarie, ben venga l'interazione delle azioni nazionali con la pianificazione regionale. Al Dipartimento della Protezione civile è affidata la ricognizione e valutazione anche degli strumenti innovativi e qui mi fermo al tema della formazione della formazione per estendere la protezione, la salvaguardia e il salvataggio anche degli animali in difficoltà. Il decreto inasprisce le sanzioni e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti. Si tratta di sanzioni amministrative e di sanzioni penali, ma nel corso dell'analisi del provvedimento in Commissione ambiente ci siamo resi conto come Forza Italia di un'anomalia che forse era sfuggita ma che per noi risultava inaccettabile: l'introduzione di una specifica aggravante generica, con aumento delle pene detentive, nell'ipotesi in cui ad appiccare il fuoco fosse chi avrebbe proprio il compito di tutelare il territorio. Abbiamo quindi condiviso con il Governo e in particolare con il Ministero della giustizia nella persona del sottosegretario Sisto, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata, l'opportunità di eliminare l'aggravante ritenendola lesiva dell'onorabilità di sindaci e operatori della Protezione civile. Appariva di fatto sproporzionata un'aggravante rispetto all'ambito di applicazione riferita alle responsabilità pubbliche che già soggiacciono a previste sanzioni,

Come bene ha ricordato la senatrice Caligiuri nel corso del suo intervento, in Italia la superficie boschiva rappresenta l'83 per cento della superficie forestale complessiva del Paese e ricopre il 29 per cento dell'intero territorio nazionale, un patrimonio inestimabile in termini di biodiversità e di ecosistemi, che però gode del triste primato, come ho ricordato all'inizio, di essere il Paese del Mediterraneo e d'Europa in cui bruciano più boschi, in particolare nelle Regioni del Sud Italia, un dato molto triste. Puglia (in particolare Sardegna, Molise, Basilicata e Abruzzo sono Regioni che vanno tutelate. In Abruzzo, poi, addirittura c'è un sistema culturale

tutelate. Concludo ricordando per l'ultima volta l'importanza dei percorsi di formazione che educhino al rispetto e al corretto smaltimento degli sfalci, delle potature e dei rifiuti in generale per evitare azioni dannose che vanno ad aggiungersi alle calamità naturali perché l'ignoranza o i paraocchi ideologici nel 2021 non possono e non devono più trovare giustificazione alcuna. Il provvedimento è per noi anche l'occasione per ribadire la posizione e la linea di Forza Italia rispetto al tema della tutela e della sostenibilità ambientale, che ci vede impegnati a dare il nostro contributo alla transizione ecologica nella maniera razionale, competente ed equilibrata che ci connota. Siamo felici che ben 14 siano i nostri emendamenti approvati, più due ordini del giorno molto importanti per le Regioni del Sud che citavo prima. convinta che per garantire tutela dell'ambiente e benessere la sostenibilità debba essere a tutto tondo (ambientale, sociale ed economica) e che questo perfetto connubio si possa realizzare solo attraverso la grande alleanza tra pubblico e privato, attraverso le riconversioni e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, che può essere governata solo attraverso un sistema strutturale della formazione a ogni livello. Prestiamo attenzione agli animali, come dimostrano molti nostri emendamenti approvati sulla necessità di estendere l'attenzione alla fauna domestica e non al loro salvataggio. Allo stesso tempo attenzione al mondo agricolo, che non può subire, oltre al danno degli incendi, anche quello della devastazione degli ungulati. Concludo dichiarando il voto favorevole di Forza Italia, approfittando dell'occasione per ringraziare i miei colleghi della Commissione ambiente, le senatrici Papatheu e Caligiuri, il senatore Messina e del prezioso ausilio i senatori Pagano e Floris; per ringraziare con tutto il cuore ogni singolo operatore, ogni singolo volontario, ogni singolo carabiniere forestale e ogni singolo vigile del fuoco per la grande opera quotidiana di altruismo e per promettere alla Sicilia, colpita ancora oggi dopo il fuoco dall'acqua, tutto il nostro impegno a dimostrazione concreta della nostra vicinanza.

approvato un decreto che oggi noi convertiamo e che pone rimedio - lo dobbiamo dire - alla vergogna di non averlo fatto prima di fronte alla piaga degli incendi che colpisce da anni

non di maniera va alla presidente Moronese e al collega Quarto. Mi fa piacere averli accanto. È stato un trio quantomeno inusuale e atipico, maggioranza e opposizione, che includeva le due anime della maggioranza forse più distanti. Aver mantenuto sempre un filo di correttezza personale ancor prima che istituzionale e politico fra noi e con il Governo penso possa essere di buon auspicio per tutti e penso possa aver contribuito - speriamo - con i nostri limiti e le nostre mancanze ad aver conseguito un risultato importante. Un ringraziamento vorrei farlo a tutti i colleghi. solo a quelli della Commissione ambiente e in parte a quelli della Commissione agricoltura, che hanno seguito con particolare attenzione il provvedimento, ma a tutti i colleghi dei territori particolarmente colpiti dagli incendi di quest'estate che, durante le audizioni, con un emendamento o capitando in Commissione per la prima volta, hanno veramente seguito il provvedimento in maniera omogenea, organica e corale, al di

e anche la migliore risposta a chi ha voluto definire quest'atto, nel migliore dei casi, un pannicello caldo. Esso è molto di più, anche per lo spirito con cui è stato assunto.

guarda all'emergenza e dall'altro ha saputo guardare alla prevenzione (e non sempre questo accade). Diciamo che il nostro è un Paese che dà il meglio di sé nell'emergenza, qualche volta solo in quel momento e magari senza saper guardare oltre. Abbiamo saputo interpretare, come Parlamento, quel ruolo che spesso rivendichiamo, ma che non sempre sappiamo portare avanti insieme. Nelle audizioni torno su questo passaggio, perché lo ritengo importante - ad andare oltre l'aspetto ideologico e a consultare non soltanto le istituzioni e le Forze dell'ordine, ma anche gli enti e le università, per avere quelle informazioni fondamentali che consentono al decisore politico di assumere iniziative e legiferare con

le associazioni di categoria degli agricoltori e la cabina di regia delle associazioni venatorie. Aver sentito tutti e aver ascoltato il punto di vista di coloro i quali subiscono comunque un danno dagli incendi, oltre ovviamente alle comunità, penso sia stato un segnale importante, che ci ha portato ad agire sul piano delle regole,

Un piano triennale con revisioni annuali permette di avere una visione complessiva; esso non solo favorisce il sostegno e la leale collaborazione fra le istituzioni, ma prevede anche giustamente, quando qualcosa non funziona, un potere sostitutivo nei confronti di quei Comuni (che sono centinaia e centinaia in Italia) che con ritardo votano in Consiglio comunale il catasto dei terreni percorsi dal fuoco. Si prevede anche che le Regioni possano agire, in caso di emergenza, riducendo i tempi. Abbiamo lottato per ogni singolo giorno, con il collega Quarto e con molti dei colleghi, e siamo arrivati a quarantacinque giorni per la perimetrazione. Avremmo voluto tutti - e dico tutti veramente - che fosse stato da subito. Speriamo che con le nuove tecnologie si possa ulteriormente ridurre

nella direzione della prevenzione e di favorire quello che nel nostro Paese funziona e che troppo spesso non mettiamo in evidenza. Dicevamo dell'organizzazione: mettere insieme tutte le forze possibili e anche veder presenti nei vari comitati soggetti provenienti da vari ambiti e da varie realtà è un aspetto fondamentale. Permettetemi di rivendicare quello che è stato un mio pallino (chiedo scusa se su questo ho insistito fino allo spasimo): la costituzione del SAVA, il Sistema aereo di vigilanza antincendio. Poter inserire coinvolgere senza spese aggiuntive il sistema, mettere in rete delle aviosuperfici e delle idrosuperfici, poter realizzare ulteriori vasche e sistemi idrici che permettono di avere i mezzi più presenti sul fronte dell'incendio, riducendo i tempi di percorrenza, coinvolgere inoltre tantissime realtà

unità di personale, la riduzione a cinque settimane del corso per i capisquadra, per poter avere persone che diano braccia e gambe a quello che abbiamo previsto nel decreto, che altrimenti rimarrebbe lettera morta. Tutti - mi auguro - speravamo di vedere di più anche con l'intervento sulle regole per la graduatoria dei discontinui, che - fa male sapere - in alcuni casi vede figurare persone per le quali abbiamo anche inasprito le pene, che dovrebbero tutelare e difendere gli incendi e invece li vanno

dalle posizioni più estreme, che magari potrebbe portarci a trovare una soluzione condivisa. Concludo con un ultimo passaggio. Quasi tutti hanno ricordato le immagini di quest'estate. Io voglio invece ricordarne altre, che sono quelle di questi ultimi giorni relative al disastro

Signor Presidente, colleghi e colleghe, membri del Governo, in queste ore il maltempo sta flagellando la Sicilia orientale e purtroppo dobbiamo registrare anche delle vittime. Tutto il MoVimento 5 Stelle si stringe intorno alle famiglie delle popolazioni colpite da questa terribile alluvione.

Quella passata è stata un'estate che difficilmente dimenticheremo. Il Paese è andato a fuoco come mai in precedenza e migliaia di ettari di verde sono andati distrutti, così come allevamenti, aziende agricole, abitazioni e animali selvatici che abitano quei luoghi. Nonostante questa tragedia, tra di noi c'è chi, come la Lega, fa giochetti senza scrupoli sulla pelle del Paese per tutelare interessi di pochi e portare acqua al proprio mulino. Piuttosto che tutelare la flora e la fauna del nostro Paese, si è preferito montare un caso su un emendamento che aveva come *ratio* semplicemente quella di sospendere l'attività venatoria per una sola stagione e solo in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza. una norma di buon senso, in quanto le fiamme hanno distrutto gli *habitat* di tantissime specie animali.

si fa comunque caccia di animali selvatici. Pertanto, questo emendamento era alquanto pertinente. Ma andiamo avanti, perché questo provvedimento è troppo importante e deve sanare una profonda ferita causata dagli incendi. Sì, perché il provvedimento in esame oggi rimedia ad una situazione gravissima, figlia di una politica miope e senza scrupoli, che non ha voluto puntare per decenni su controllo e prevenzione; la stessa politica che ha cancellato quella risorsa preziosissima rappresentata dal Corpo forestale dello Stato (e anche qui le colpe hanno un nome e un cognome). E così ogni anno migliaia di incendi hanno devastato e distrutto migliaia di ettari di bosco, gli stessi boschi che dovrebbero catturare la CO₂ e aiutare i nostri territori a depurare l'aria e a combattere il cambiamento climatico. A ricordare i drammi del passato ci pensa Ferdinando Cotugno, giornalista e scrittore, nel suo libro «Italian woood». Negli ultimi decenni, i roghi boschivi sono stati un'emergenza nazionale. Il 2017 fu un anno terribile: secondo i dati dei Vigili del fuoco, ci fu un incremento del 321,6 per cento, con particolare sofferenza delle aree più calde, il Sud e le isole. Tra il 2009 e il 2016 un ettaro su tre è andato in fumo in Sicilia, uno su cinque in Sardegna. Nel 2018 c'è stato un calo del 90 per cento, con una ripresa dei roghi nel 2019. Negli ultimi trent'anni, secondo i dati della Protezione civile, è andato distrutto a causa delle fiamme il 12 per cento del patrimonio forestale nazionale. Tra il 1980 e il 2009 - ricorda Cotugno - la superficie media incendiata per anno era di 111.665 ettari.

Gli incendi di quest'anno hanno superato il *record* del 2017. Secondo l'ultimo inventario forestale, in Italia si contano oggi ben 11 milioni di ettari, cioè il 36,7 per cento del territorio da Nord a Sud: più di un terzo dell'Italia, una grande responsabilità che il nostro Paese non ha ancora accettato. In Sicilia, da cui sono arrivate le immagini terrificanti e dove le fiamme hanno divorato oasi bellissime, pare siano stati bruciati circa 80.000 ettari, pari al 3 per cento della Regione. In Sardegna, dove sono andati a fuoco oltre 20.000 ettari di boschi, secondo stime della Coldiretti ci vorranno almeno quindici anni per ripristinare la flora e la fauna. I danni sono ingenti, come per tutto il Paese, con un costo calcolato di circa 1 miliardo di euro, tra opere di spegnimento, di bonifica e di ricostruzione a livello nazionale. Con questo decreto-legge oggi poniamo le basi per affrontare il problema degli incendi da qui ai prossimi anni. Sia chiaro, questo rappresenta un primo passo; toccherà fare di più nei prossimi mesi con il lavoro parlamentare, soprattutto a supporto delle Regioni, il cui lavoro in questi anni a tutela dei nostri boschi è stato a dir poco carente. Detto questo, ora bisogna guardare al futuro, auspicando che alcuni errori non vengano commessi nuovamente. Questo decreto-legge rafforza notevolmente il Dipartimento della protezione civile ha proprio come obiettivo quello di stilare con cadenza triennale il Piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri, necessarie per una più adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; un documento che andrà a integrare la consueta pianificazione regionale. Il decreto-legge esame dà ampia importanza al ruolo delle tecnologie e di tutti quegli strumenti atti al monitoraggio dei nostri territori. Mezzi, ma soprattutto formazione, perché è principalmente sulla formazione che dobbiamo puntare. Auspico vivamente che nei prossimi mesi, partendo dalla legge di bilancio, si possa ampliare lo spettro di interventi a favore della prevenzione dei nostri territori. L'Italia è un Paese fragile; non lo scopriamo oggi. È noto quanto costi meno la prevenzione rispetto alla riparazione dei danni di temporali e incendi. Si parta allora da ciò che è necessario per questa terra. Sono questi i temi che dobbiamo approfondire nel 2021, che attende alla finestra il 2022.

Partiamo dal decreto-legge incendi avendo come visione un quadro più ampio. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento

Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi della Commissione per il risultato ottenuto con il più ampio consenso. Si tratta di un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare, modificato in sede emendativa nel corso dell'esame in Commissione, volto a introdurre un nuovo comma all'articolo 119 della Costituzione, con il quale si esplicita il concetto che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Più nello specifico la Costituzione del 1948 contemplava, al terzo comma, dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerata la realtà svantaggiata sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione. Si stabiliva infatti che «per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali». Con la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, avvenuta nel 2001, è stato eliminato ogni richiamo all'insularità dal dettato costituzionale, permanendo soltanto un riferimento ai territori con minore capacità fiscale per abitante a prescindere dalle condizioni geografiche. Con le modifiche introdotte all'articolo 119 è stato inserito inoltre il principio del federalismo fiscale con l'obiettivo di creare uno stretto legame tra decisioni di spesa e di prelievo, diretto ad avvicinare i cittadini alle istituzioni, nel senso di favorire un'allocazione delle risorse pubbliche in termini di beni e servizi più rispondenti alle preferenze di coloro che sono chiamati a sostenerne il costo. Alla luce dell'articolato ciclo di audizioni informali di costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di associazioni e comitati, sono state apportate delle modificazioni al testo originario con l'obiettivo di evitare, ad esempio, che il termine insularità in Costituzione sia considerato solo come una mera fonte di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario. Per tale ragione è stato inserito il riferimento al riconoscimento delle peculiarità delle isole, espressione che se intesa in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle specialità e non ad una mera presa d'atto, sottende una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori. Pertanto la Repubblica, che riconosce la particolare natura delle isole, si impegna a promuovere tutte le misure necessarie a valorizzare le peculiarità ed evitare che le stesse possano diventare fonte di svantaggi per i medesimi territori. Si rafforza ancora di più, con questa riforma, il concetto che non basta la realizzazione di fondi perequativi senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante, ma serve un atteggiamento non più volto esclusivamente al riequilibrio di sbilanciamenti esistenti, ma propositivo, nell'ottica dell'esaltazione delle peculiarità territoriali. Pertanto, Presidente, auspico che quest'Assemblea si esprima all'unisono sul contenuto della proposta al nostro esame. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà. Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il disegno di legge costituzionale oggi in discussione è frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione affari costituzionali in Senato, e colgo anzi l'occasione proprio per ringraziare il relatore Garruti per il risultato che si è riusciti a raggiungere. Si tratta di un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare, modificato in sede emendativa nel corso dell'esame in Commissione, volto a introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Alla luce dell'articolato ciclo di audizioni informali di costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari, esponenti di associazioni e comitati, sono infatti state apportate modificazioni al testo originario, con l'obiettivo di evitare che il termine «insularità» in Costituzione sia considerato una mera fonte di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario. Per questa ragione, essendo tra l'altro sarda conoscendo in prima persona le particolarità di un territorio così geograficamente eterogeneo e singolare, ma strettamente legato alla propria storia, è stato inserito un riferimento al riconoscimento della peculiarità delle isole, espressione che, se intesa in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle specificità, e non legata a una mera presa d'atto, sottende a una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori. Più nello specifico, la Costituzione del 1948 contemplava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento all'insularità: le isole, percepite come realtà svantaggiate dal punto di vista geografico, economico e sociale, erano infatti destinatarie di contributi speciali da parte dello Stato centrale. Tuttavia, con la riforma del Titolo V, avvenuta nel 2001, tale riferimento costituzionale è stato eliminato e, con la modifica all'articolo 119, è stato inserito il principio del federalismo fiscale, con l'obiettivo di creare uno stretto legame tra le decisioni di spesa e di prelievo diretto ad avvicinare i cittadini alle istituzioni, nel senso di favorire un'allocazione delle risorse pubbliche in termini di beni e servizi più rispondenti alle preferenze di coloro che sono chiamati a sostenerne il costo. Il processo di attuazione dell'articolo 119 ha preso avvio con la legge delega del 2009, approvata, quindi, a distanza di circa otto anni dalla riforma costituzionale del Titolo V, che ha portato il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi delegati e che recava - tra i principi e i criteri direttivi - la necessità di tener conto delle specificità delle realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani, alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale. Il riconoscimento dell'esigenza di un intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità è contenuto anche in interventi legislativi successivi alla legge n. 42 del 2009, che sono stati diretti a specifiche realtà insulari quali la Sicilia e la Sardegna e non al complesso delle isole italiane. Mi riferisco, ad esempio, all'attribuzione di fondi alla Sardegna per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e che assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, così come previsto dal decreto-legge n. 185 del 2015. Penso anche all'istituzione di un comitato istruttore paritetico tra Stato e Regione nella legge di bilancio del 2018, per l'attuazione della procedura di riconoscimento alla Sardegna dello *status* di Regione insulare, fnalizzato alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le Regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea, individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a cui sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati. Inoltre la legge di bilancio del 2020 è intervenuta nell'ambito del recepimento dell'accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo e la Regione Sardegna, rinviando ad una sede *ad hoc* la definizione della questione della compensazione dei costi dell'insularità.

che attribuisce al comma 4 dell'articolo 14 finanziamenti da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. È un dato di fatto che le isole presentino intrinseche situazioni di svantaggio, che riguardano i trasporti e la connessione con la terraferma, l'ambiente e diversi ecosistemi fragili, esposti a costanti cambiamenti climatici, oppure la ridotta attività economica, comprensiva di turismo stagionale, pesca e agricoltura. però al contempo impossibile negare il loro ruolo essenziale, leva per l'economia e la storia del nostro Paese. In altri termini, data l'incidenza della condizione di insularità nello sviluppo di territori strategici come Sardegna e Sicilia,

diversi comitati di cittadini il 7 aprile 2018 hanno iniziato il processo di raccolta firme, volto a favorire la presentazione, all'interno del Parlamento italiano, di un disegno di legge costituzionale finalizzato a riportare il tema dell'insularità e delle pari opportunità dei cittadini residenti nelle isole al centro del dibattito nazionale. È un invito che dobbiamo accettare tutti, oggi, in questa Assemblea e che io stessa ho fatto mio, proprio per le mie origini sarde, anche con la presentazione di un disegno di legge a mia prima firma, volto ad istituire, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la circoscrizione elettorale della Sardegna. Signor Presidente, concludo che oggi dobbiamo ripartire dal riconoscimento effettivo della condizione di insularità, che deve passare dalla previsione costituzionale, per poi arrivare all'applicazione pratica delle politiche dell'Unione europea e di quelle nazionali. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

subisce, sia quando si traghetta, sia quando si passa con la macchina. E questo quando va bene, perché poi, anche dal punto di vista degli investimenti in queste infrastrutture, è tutto un punto interrogativo. Alle volte le navi che ci devono portare sono ferme, altre volte sono insufficienti, come in

non possono prendere mezzi inevitabilmente legati a spostamenti di treno, aereo o macchina, soprattutto oggi che il costo della benzina è ancora aumentato. Vi ricordo che il mio biglietto ferroviario, per esempio di un vagone cuccetta, costa dai 150 ai 200 euro e io viaggio spesso anche in seconda classe, perché non c'è posto (anche questo è un altro problema, dovendoci tutti trasferire con i treni o con i mezzi). Sugli aerei, peggio mi sento. Vedrete che durante tutto il periodo delle feste natalizie i più fortunati riusciranno a trovare un biglietto da 500, 400, 600 euro su questo ovviamente invito tutti a una riflessione. Il problema dell'insularità non può essere risolto sempre demandandolo ai Governi, con la richiesta di risorse economiche volte a colmare questo *gap*. Noi dobbiamo puntare al riconoscimento dell'insularità dell'insularità come condizione e prerequisito di sviluppo, soprattutto per sanare la competitività di queste Regioni rispetto ad altre. E questi sono i trasporti che vivo io, da pendolare;

Infatti, con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, approvata nel 2001, è stato soppresso il terzo comma dell'articolo 119, che prevedeva contributi speciali per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Si trattava di una norma voluta dai Padri costituenti per garantire l'unità territoriale e la coesione sociale, attraverso la tutela speciale di alcune aree del Paese economicamente più svantaggiate in ragione della loro collocazione geografica. Il riconoscimento dello svantaggio territoriale nasceva dalla volontà di garantire a tutti i cittadini italiani, ovunque fossero residenti, un'eguale prospettiva nel processo di crescita complessiva, in campo economico, sociale e culturale, fattori determinanti per lo sviluppo e per il futuro del Paese. Il legislatore intendeva, quindi, favorire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona e della collettività. È la stessa richiesta che oggi, attraverso il disegno di legge costituzionale all'esame dell'Assemblea del Senato, ci viene sollecitata da centinaia di migliaia di nostri cittadini. L'Assemblea costituente aveva ben presente, come sottolineato da Benedetto Croce, che le questioni meridionali *post* risorgimentali erano ancora aperte. Si riconobbe, infatti, lo statuto speciale per le isole maggiori ed interventi mirati, come quelli poi sostenuti dalla Cassa del Mezzogiorno. Lo Stato intendeva conciliare compiutamente l'unità territoriale e l'autonomia. purtroppo è venuta meno la questione dell'insularità ed è significativo il fatto che più di 200.000 cittadini, su tutto il territorio nazionale, si siano mobilitati per sottoscrivere e presentare alle Camere una proposta di legge costituzionale affinché la Repubblica italiana riconosca gli svantaggi strutturali derivanti dall'insularità e adotti le misure necessarie necessarie per rimuoverli. Il riferimento all'insularità ovviamente non riguarda solamente la Sicilia e la Sardegna, ma si estende anche alle isole minori. In buona sostanza, colleghi, centinaia di migliaia di nostri concittadini non soltanto quelli che vivono nelle splendide isole italiane - hanno rivelato al corpo legislativo gli svantaggi e le criticità propri di questa discontinuità territoriale, svantaggi che impediscono il godimento uniforme delle prestazioni dei diritti civili e sociali che sono propri della cittadinanza. Vorrei evidenziare la circostanza che, dopo la Brexit, l'Italia è diventato il Paese europeo in cui risiede la maggior parte dei cittadini insulari: il 12 per cento della popolazione. L'ambizioso progetto di operare una ricognizione delle infrastrutture insulari, previsto dalla legge delega in materia di federalismo fiscale nel 2009 - la legge che a distanza di otto anni ha avviato un processo di attuazione della riforma dell'articolo 119 del Titolo V, in base al quale si sarebbero dovuti programmare interventi mirati per strutture sanitarie, scuole, reti stradali, autostrade, ferrovie, reti idriche, elettriche e di trasporto, distribuzione del gas, strutture portuali e aeroportuali - ancora non ha avuto piena attuazione. In conseguenza di ciò, i contributi mirati, con cui si dovrebbero finanziare i programmi pluriennali per gli interventi, non sono stati quantificati in modo congruo. La formulazione del terzo comma dell'articolo 119, nella sua versione originaria, per taluni aspetti era analoga a quella del comma che il disegno di legge costituzionale al nostro esame vorrebbe aggiungere allo stesso articolo 119, reintroducendo il riferimento alla valorizzazione delle isole come finalità prioritaria dell'intervento statale. Tale riconoscimento verrebbe a costituire per i legislatori un vincolo da rispettare. Anche l'ordinamento dell'Unione europea prevede che alle Regioni ultraperiferiche possano essere destinati aiuti da parte degli Stati per superare la persistenza di tutti questi fattori che, sommati, recano un grave danno allo sviluppo del territorio. Si pensi alle misure per favorire la continuità territoriale, riconosciuta dalla stessa Unione europea come presupposto del diritto fondamentale di libertà di circolazione e di soggiorno. Da tempo la Regione Sicilia ha chiesto al Governo interventi concreti per garantire ai siciliani il diritto alla continuità territoriale e superare gli svantaggi competitivi strutturali e permanenti che tale discontinuità comporta, tale discontinuità comporta, anche se - colleghi - confido che, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate, tale divario possa essere finalmente colmato; continuità territoriale a cui dobbiamo pensare anche in termini di attività di circolazione delle merci, che può essere compromessa da un'offerta insufficiente di servizi di trasporto. La politica deve far sì che anche nei territori insulari siano favoriti lo sviluppo, l'insediamento di imprese e la realizzazione di infrastrutture moderne. È anche per questo che guardo con fiducia al PNRR.

È iscritto a parlare il senatore Doria. Ne ha facoltà. è per me un momento di grande soddisfazione, in cui viene riconosciuto quanto per decenni è stato oggetto di battaglie da parte di chi mi ha preceduto, con l'obiettivo di perseguire quella felicità dei sardi che anche lo statuto del Partito Sardo d'Azione annovera da sempre tra i suoi obiettivi principali. un partito che quest'anno ha compiuto cent'anni dalla sua nascita, che ha sempre sostenuto le battaglie autonomiste e identitarie, condividendo oggi con la Lega lo spirito federalista di sempre. La Sardegna è un'isola fiera della sua cultura e storia millenaria, ma anche limitata nel suo sviluppo economico, oggi più di ieri, da quel *gap* rappresentato dall'insularità. Questa, se da un punto di vista filogenetico ha favorito le alchimie genomiche, che hanno fatto della Sardegna la terra dei centenari famosa in tutto il mondo, dall'altra ha determinato un'inaccettabile disparità nello sviluppo socioeconomico che va oggi colmata. Tutte le isole, chi più chi meno, presentano situazioni di svantaggio che riguardano vari ambiti, primi fra tutti i trasporti e l'ambiente. In tema di trasporti, alla Sardegna occorre una vera continuità territoriale marittima ed aerea, duratura nel tempo e non legata a scadenze e proroghe che generano incertezze e diseconomie. La Sardegna, Regione a vocazione turistica, ha iniziato a vedere uno spiraglio di ripresa economica dopo il disastro determinato dalla pandemia e non ha certo bisogno dell'incertezza legata a un sistema di trasporti costoso, inadeguato e penalizzante. Se è un dato inequivocabile il diritto dei sardi alla mobilità da e per la Sardegna al pari del resto degli italiani che vivono e si muovono nella Penisola, non da meno deve essere garantito il diritto a una continuità per le merci in entrata e in uscita dall'isola, che ridurrebbe il *gap* derivante dal costo dell'insularità, eterna palla al piede di chi decide di fare impresa in Sardegna. A tal fine abbiamo più volte richiesto ai vari Governi che si sono succeduti nel tempo una nuova continuità territoriale che abbatta i costi di trasporto per persone e merci, ma anche un sistema di trasporto con elevati *standard* di qualità che siano degni di un Paese civile. L'affidamento ai vettori delle rotte in continuità territoriale può reggersi, infatti, non solo con il criterio del basso costo, ma piuttosto su un'offerta complessiva che miri alla qualità del servizio, frequenza dei servizi e maggiori rotte. La qualità e il *comfort* offerto dai traghetti che solcano le rotte per la Sardegna e la Penisola devono servire come biglietto da visita del nostro comparto turistico e come primo giorno di vacanza per chi decide di trascorrere le ferie nella nostra terra. Tuttavia, se la continuità marittima piange, quella aerea di certo non ride. continuità aerea imposta alla Sardegna da Roma e da Bruxelles ha concesso di connettere i tre aeroporti sardi con i soli *hub* di Linate e Fiumicino. Ma, per una libera circolazione dei passeggeri e delle merci, con ovvio rilancio dell'economia, sarebbe invece necessario collegare i tre aeroporti principali sardi anche con gli aeroporti di altre realtà realtà produttive del Paese. Da anni, però, il bando è bloccato al vaglio della Commissione europea, a causa di un'incomprensibile ipotesi di violazione delle regole del mercato che valgono per noi, ma non per la Corsica. Dopo il suo insediamento, il presidente della Regione Christian Solinas, già membro di quest'Assemblea, in una situazione incerta per il mancato rinnovo del bando di continuità aerea fermo Bruxelles, ha dovuto affrontare uno dei più grandi *crack* economico-finanziari della storia dell'aviazione civile italiana, con il fallimento di Air Italy che, oltre ad aver messo sulla strada 1.500 dipendenti specializzati e le loro famiglie, ha anche lasciato il monopolio delle rotte ad Alitalia, che nei giorni scorsi ci ha salutato per sempre, travolgendoci fra scioperi e disservizi. Oggi si viaggia con Volotea, vettore *low cost* spagnolo, che assicurerà il servizio fino a maggio e poi non è dato saperlo. Viene proprio da dire che del domani non c'è certezza e lo sviluppo economico di un'isola non si può certo basare su questi presupposti. In tema di ambiente, le isole sono state spesso caratterizzate da un ecosistema fragile, particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l'erosione della costa, la siccità e la scarsità di risorse naturali, che si collega alla dipendenza energetica con la terraferma. Tale situazione suggerisce un intervento pubblico per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in generale, l'adozione delle misure volte alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Alla luce di queste considerazioni oggi plaudo al disegno di legge costituzionale n. 865, d'iniziativa popolare, che mira a riconoscere il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e introduce un comma aggiuntivo dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in cui solennemente la Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. La disposizione pone in capo alla Repubblica il compito di riconoscere la situazione di svantaggio e di provvedere alle necessarie misure attraverso l'individuazione delle relative risorse necessarie. Per apprezzare la portata innovativa del disegno di legge in esame, desidero richiamare i contenuti dell'articolo 119 della Costituzione e in particolare il quinto comma, a cui si ricollega il provvedimento da un punto di vista contenutistico. In estrema sintesi, le modifiche all'articolo 119 introdotte nel 2001 hanno inserito l'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali in quello che conosciamo come federalismo fiscale, corredata da un duplice sistema perequativo. Il quinto comma dispone in ordine a risorse statali aggiuntive nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione, da parte dello Stato, di interventi speciali in favore di tali enti, al fine di perseguire le seguenti finalità: promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Per un più efficace inquadramento del disegno di legge costituzionale in esame può essere di ausilio sottolineare, purtroppo, lo stato di parziale attuazione dell'articolo 119, che potrebbe aiutare a comprendere le ragioni di coloro che rilevano l'inadeguatezza del sostegno ai territori con vantaggi strutturali, tra i quali possono essere compresi quelli insulari. L'articolo 119 prevede un sistema in cui l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa si collega a un duplice sistema perequativo: un primo senza vincolo di destinazione in favore degli enti territoriali con minore capacità fiscale per abitante, che è stato interpretato in sede attuativa come riferito a supportare le funzioni ordinarie degli enti territoriali; un secondo di carattere strutturale per scopi diversi rispetto all'esercizio normale delle funzioni. In questo quadro, una completa attuazione dell'articolo 119, avrebbe potuto assicurare interventi mirati a contrastare lo svantaggio naturale dei territori insulari e garantire un'effettiva parità con i cittadini della terraferma nel godimento dei diritti individuali inalienabili. Oggi, con la modifica all'articolo 119, attraverso l'introduzione del nuovo comma più stringente, vogliamo solennemente sottolineare come il principio di insularità introdotto voglia tutelare i diritti di tanti italiani che non possono essere più calpestati ed è per questo che oggi con fiducia vi invito a sostenere questo disegno di legge.

proprio questa mattina, dalle pagine della «Nuova Sardegna», abbiamo appreso della notizia di una signora cinquantenne di Olbia che, costretta per un delicato intervento chirurgico a operarsi nel Nord Italia, ha riscontrato che l'unico mezzo disponibile per tornare ad Olbia in barella fosse la aeroambulanza. È stata così costretta a spendere quasi 10.000 euro per tornare a casa dalla sua famiglia. Le condizioni di salute di questa signora non le permettono di affrontare un lungo viaggio in mare. Inoltre, la compagnia aerea, a cui alcuni giorni fa sono state assegnate le rotte in continuità territoriale, ancora non fornisce servizi per i cittadini in barella, che sono spesso costretti ad andare in altre Regioni per sottoporsi a interventi chirurgici complicati, vista anche la difficile situazione sanitaria che stiamo vivendo proprio negli ultimi giorni in Sardegna. Questo è un esempio plastico e tangibile di cosa può significare vivere in un'isola. Oggi siamo chiamati a esaminare un provvedimento molto importante e atteso da tanto tempo per il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità. Nel nostro Paese le isole sono oltre 800, di cui un'ottantina abitate e i cui residenti si trovano da sempre in una situazione oggettiva di diversità e di svantaggio rispetto al resto d'Italia. È pertanto necessario garantire loro una effettiva parità nel godimento e nel rispetto dei diritti previsti dalla nostra Costituzione. Agli svantaggi che quotidianamente sono costretti a vivere i cittadini sardi e i cittadini isolani aggiungiamo, con il resto d'Italia e d'Europa, anche la mancanza di pari opportunità occupazionali, infrastrutturali, di sviluppo economico e di benessere. In Sardegna - ad esempio - occorre sviluppare e dare impulso a infrastrutture di qualità affidabili e sostenibili. Penso in particolare ai servizi ferroviari spesso obsoleti e con tempi di percorrenza troppo lunghi e nessun investimento significativo in vista. Occorre anche sostenere lo sviluppo economico attraverso l'istituzione della ZES, una zona dotata di una legislazione economica di svantaggio di grande rilevanza, in virtù anche di numerosi benefici fiscali e delle misure di semplificazione previste che possono rappresentare un volano per la nostra economia, che paga un prezzo ancora troppo alto proprio per la sua insularità; svantaggio particolarmente evidente in un'epoca come quella attuale di forte interdipendenza geografica ed economica. Proprio perché l'insularità condiziona spesso negativamente tutti gli aspetti della vita quotidiana dei propri cittadini, è necessario e urgente dare alle nostre isole un tangibile riconoscimento istituzionale e costituzionale. Lo Stato deve garantire pieni diritti e opportunità ai milioni di cittadini che abitano, studiano, lavorano e investono nelle nostre isole, ricordando sempre che queste persone sono costrette a convivere con tanti disservizi a cui fanno fronte con coraggio e determinazione. determinazione. Ritengo che quindi il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare che ci apprestiamo ad approvare e che auspico trovi il consenso di tutti i colleghi oggi in quest'Aula vada nella giusta direzione. E ringrazio per questo risultato il comitato che ha promosso il disegno di legge e tutti i colleghi senatori sardi che non si sono risparmiati nel portare avanti, anche all'interno dei propri Gruppi, la stessa proposta. Sia, quindi, data piena dignità costituzionale alle nostre meravigliose isole, affidando allo Stato il compito di rimuovere i troppi ostacoli che ancora condizionano la vita degli isolani. *(Applausi)*.

di posticipare alla prossima settimana la replica dei relatori, le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento.

Signor Presidente, il disegno di legge sui titoli universitari abilitanti, approvato in prima lettura alla Camera e che ha superato senza modifiche l'esame della Commissione istruzione al Senato, figura tra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che devono ottenere il via libera entro il 31 dicembre prossimo. Il provvedimento attribuisce effetto abilitante ad alcune lauree ai fini dell'esercizio delle rispettive professioni. Nello specifico, l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria, nonché della laurea magistrale in psicologia, abilita all'esercizio delle professioni rispettivamente di odontoiatria, farmacista, medico veterinario e psicologo. Analogamente il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e professioni tecniche industriali e dell'informazione ha effetto abilitante all'esercizio della professione di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. Inoltre, il possesso delle lauree magistrali in chimica fisica e biologia abilita rispettivamente all'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologico. Oltre alle menzionate lauree, il disegno di legge prevede che, con regolamenti di delegificazione, e quindi non più con legge, si possono rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate ulteriori lauree. Si tratta di un intervento organico con cui si estende ad altri ambiti professionali la misura avviata con l'articolo 102 del decreto cura Italia, che ha introdotto la laurea abilitante in medicina e chirurgia, consentendo di fornire una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale in seguito all'emergenza pandemica. Ulteriori integrazioni saranno possibili al tavolo che il Governo si è impegnato ad attivare in tempi celeri per la revisione e l'aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, dando seguito alle istanze provenienti da alcune professioni in un'ottica di completamento del quadro normativo di riferimento. La legge non comporterà scavalcamenti, in quanto il dispositivo abilitante alla professione decorrerà non dall'entrata in vigore della norma, bensì dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, previo accreditamento dei corsi di studio abilitanti. Costituisce un primo tassello cui faranno seguito disposizioni attuative del Governo e delle università e la fase di accreditamento. Coloro che hanno già conseguito il titolo in base ai previgenti ordinamenti didattici, o lo conseguiranno nel frattempo, per accedere alle rispettive professioni dovranno sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione. Tuttavia, l'articolo 6 dispone che siano assicurate modalità semplificate. La loro definizione sarà rimessa a uno o più decreti del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio. Per gli studenti che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, è prevista una specifica disciplina transitoria (articolo 7). L'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sarà acquisita previo superamento di un tirocinio pratico valutativo e di una prova pratica valutativa. Anche in questo caso la disciplina concreta è rimessa al decreto del Ministro dell'università.

L'altro ordine del giorno riguarda invece la figura dell'assistente sociale. L'emendamento in esame viene un po' a completamento e ci tengo a spiegarne il contenuto.

ragazzi e bambini all'interno dei nuclei familiari, noi dovremmo potenziare la figura dell'assistente sociale,

nel passaggio dal decreto del 1999, che prevedeva la laurea magistrale (quindi il quinquennio), al decreto ministeriale n. 270 del 2004, che ha dato vita alla suddivisione tra la laurea triennale e la laurea specialistica biennale. Sostanzialmente in questo passaggio è intervenuto un decreto interministeriale che ha equiparato alcune classi di concorso che una volta includevano la laurea conseguita in cinque anni e quella conseguita con i primi tre anni nella facoltà di scienze politiche.

affinché venga considerato l'articolo 23, permettendo ai nuovi laureandi di essere sottoposti a un esame, possibilmente da parte di personale specializzato appartenente all'albo degli assistenti sociali. Con questo tentativo

sezione B, che invece a livello internazionale si considera *in toto*. Addirittura intervengono in questa direzione in questa direzione sia le linee guida relative agli *standard* educativi approvate dall'Associazione internazionale delle scuole di servizio sociale, sia la Federazione internazionale degli assistenti sociali. Arrivo al dunque:

che al Ministero dell'interno la Divisione anticrimine, insieme al CNOAS e ad altre figure, sta stilando un protocollo di intervento nei casi di violenza anche sulle donne. È un'emergenza.

un ulteriore tassello a quella riforma nata nel pieno dell'emergenza pandemica quando, con la legge n. 18 del 2020, per far fronte alla carenza del personale medico venne introdotto il valore della laurea abilitante nell'ambito della laurea magistrale in medicina. Dopo quel positivo precedente, era doveroso che si allargasse il potere abilitante agli altri corsi dell'area medico-chirurgica per l'esercizio delle professioni di odontoiatria, farmacista, veterinario e psicologo, così come per le professioni di tecnico agrario, geometra, perito agrario e perito industriale. Allo stesso tempo, il provvedimento prevede che in questi corsi di laurea un terzo dell'attività sia dedicato alla tecnica e ben due terzi alla parte pratica. inutile sottolinearne l'importanza in un Paese in cui storicamente la formazione universitaria si è quasi sempre concentrata sulla parte teorica. Altri due elementi degni di nota sono i seguenti. In primo luogo, questo in esame non è un provvedimento chiuso ad alcuni corsi di laurea: con l'articolo 4 viene conferita la possibilità ad altri ordini professionali e alle università di poter aderire in una seconda fase, con benefici per l'università che lo fanno adeguando i regolamenti dell'ateneo stesso. Il secondo elemento positivo è l'aver scongiurato un rischio, ossia la mortificazione degli ordini professionali. Questo disegno di legge ribadisce invece la loro importanza, ne rinnova il valore fondativo rispetto a professioni che richiedono qualità, deontologia, continuo aggiornamento professionale, nonché tutela dei cittadini dalle forme di esercizio abusivo o illegittimo. davvero che questo provvedimento vada nella direzione, più volte auspicata, di ambiti professionali con meno colli di imbuto, con legame diretto, direi consequenziale, tra ottenimento di titoli di studio e l'esercizio della professione per cui si è studiato. Certo, non siamo davanti a norme che chiudono definitivamente la questione, perché - come abbiamo visto e ribadito più volte - le implicazioni sono numerose: basti pensare al grande impegno in termini di riforma che si chiede al sistema universitario. abbiamo forte bisogno di puntare con ancor maggior vigore alla formazione ad alto livello sulla ricerca, per renderla elemento strutturale del sistema Italia, come lo ha ricordato bene il premio Nobel Giorgio Parisi. La strada intrapresa con questo provvedimento, che va concretamente incontro ai nostri giovani, alle studentesse e agli studenti, è sicuramente quella giusta. Pertanto, ribadisco volentieri il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

Vorrei sottolineare l'importanza del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare oggi, proprio perché reca nuove norme che mirano a snellire e semplificare l'accesso ad alcune professioni, garantendo quindi agli studenti un accesso più rapido nel mondo del lavoro; dunque l'acquisto del titolo senza tempi di attesa, cancellando l'esame di Stato in alcune professioni proprio per garantire una maggiore concorrenza in alcuni settori. Non solo, il disegno di legge apre alla possibilità di ulteriori titoli universitari. Già questa breve introduzione sarebbe sufficiente a cogliere la rilevanza di un simile provvedimento. Ci sono però due elementi di contesto che vorrei mettere in luce. Il primo elemento è lo stretto legame tra questo provvedimento e il PNRR: si tratta proprio di un lavoro importante di correlazione tra mondo universitario e mondo del lavoro.

Già questi dati allarmano non poco e ci interrogano su una valutazione complessiva dell'attuale sistema, anche a fronte di un sistema di lavoro che ricerca figure di professionisti sempre più specializzati. Permettetemi però di ringraziare il relatore e tutte le colleghe e i colleghi della mia Commissione e di tutte le Commissioni che hanno lavorato sul testo, rivolgendo altresì un ringraziamento alla ministra Messa, che non si è limitata a ereditare un provvedimento dal precedente Esecutivo, ma ha posto le basi per un confronto in grado di ottenere i miglioramenti cui si è giunti nella fase di approvazione del provvedimento Certamente, come la Ministra sa per esserci confrontati durante la Commissione, resta il rammarico che non siano state ascoltate pienamente le istanze provenienti da altri rappresentanti della società civile, che non trovano purtroppo spazio nella legge. Il Gruppo Italia Viva-PSI ha cercato di farsi portavoce di quelle esigenze e di quelle istanze; penso - ad esempio - alla proposta che avevamo avanzato in merito alla modifica dei requisiti di accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'ordine degli assistenti sociali o alla modifica della disciplina dell'albo professionale dei biologi. Avremmo voluto maggiori margini di ascolto e di manovra, ma sono sicura - grazie anche alle parole di rassicurazione della Ministra in Commissione - che tali istanze troveranno comunque spazio in altri provvedimenti. Vorrei poi infine sottolineare che non è minimamente intaccata la preparazione dei professionisti con il provvedimento al nostro esame, proprio perché si sceglie semplicemente di anticipare a una fase prodromica l'ingresso nel lavoro, e ancora di più non solo attraverso la puntuale verifica delle competenze tecniche e pratiche proprio dei professionisti stessi.

sarebbe importante poter rendere abilitante anche questo tipo di formazione. Vorrei sottolineare anche il fatto che Fratelli d'Italia è molto attenta al mondo dei giovani, quindi a permettere l'inserimento nel mondo del lavoro quasi

perché, se notiamo, lo spostamento dell'età di una primipara rispetto al picco della fertilità per una donna - che è di venticinque anni - è dieci anni dopo, proprio in seguito al percorso di studi

hanno competenze imprescindibili come dimostrare un comportamento etico e professionale, dare valore e includere la diversità e la differenza, promuovere i diritti umani e la giustizia sociale, economica e ambientale; la valutazione, progettazione e implementazione dell'intervento sociale con individui, famiglie, gruppi, organizzazioni e comunità. Ripeto, a livello internazionale è già stata posta l'attenzione sull'importanza della figura, ma vorrei anche mettere in risalto che in questo momento, nella Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza,

con figure apicali del territorio catanese, ed è emerso come l'intervento dei servizi sociali sia importante per coordinare e come, invece, l'intervento di alcune associazioni di tutela delle donne

di completare lo studio dei tre anni. Altrimenti i laureati in scienze politiche, che hanno la loro formazione, anziché vederli, come nostri collaboratori o tra i nostri scanni, li vedremo fare gli assistenti sociali, senza averne la formazione adeguata.

li portava ad avere percorsi e tempistiche disomogenei e indubbiamente una maggiore difficoltà rispetto al resto dei loro "cugini" europei.

tra il mondo dell'università e il mondo delle professioni. Si tratta di una cosa non così scontata in Italia, che è stata sperimentata tanti anni fa e che poi era rimasta lì;

Sono contenta che questo ramo del Parlamento si trovi oggi ad affrontare, a poter votare, a rendere definitivamente legge questa opportunità per i nostri ragazzi. Sono altresì contenta che, nella prossima tabella di marcia, proprio questo ramo del Parlamento si troverà ad affrontare che rappresentano un altro tassello fondamentale per poter avvicinare i nostri ragazzi al mondo del lavoro. La ministra Messa, che vedo in

queste potranno essere recuperate quasi nell'immediato, con provvedimenti successivi che armonizzeranno tutto il sistema, mantenendo però la specificità dei percorsi che che la legge che noi oggi votiamo in questa sede garantisce e struttura, ripeto, unendo il mondo dell'università al mondo delle professioni. Vi chiedo solo di consentirmi una piccola nota di natura personale. Il Gruppo Partito Democratico già nella scorsa legislatura aveva

esisteva nel Paese e che noi volevamo rendere abilitante. Questo percorso è stato seguito, nella sua stesura in quegli anni, da una persona

sia significativa, perché un uomo che ha amato così tanto l'università, che è stato un innovatore e che ha voluto portare degli elementi nuovi nel sistema universitario, provando a essere un po' pioniere, sia anche lui parte di questo risultato che, grazie al lavoro della Ministra, del Governo e delle Commissioni, riusciamo a portare a casa. *(Applausi)*. Signor Presidente, ministro Messa, colleghi senatori, di questi giorni il confronto, piuttosto vivace, tra il Governo e i sindacati sulla riforma delle pensioni, con i sindacati che, come è noto, avendo la prevalenza dei propri iscritti tra i pensionati, difendono la categoria e cercano di anticipare il più possibile il passaggio dal mondo del lavoro alla pensione e il Governo che si preoccupa necessariamente di tenere in equilibrio il sistema previdenziale e di creare le condizioni per colmare il *gap* dell'occupazione giovanile. Sappiamo, per esperienza diretta (non che non fosse prevedibile quando la norma è stata varata), che quota 100, oltre ad aver avuto un impatto enorme sui conti pubblici (11 miliardi), non ha onorato l'impegno di creare quel vuoto di lavoratori in là negli anni perché fosse riempito in pari misura da giovani neoassunti. I dati dell'OCSE ci ricordano che la disoccupazione giovanile in Italia è superiore al 33 per Allarme nell'allarme: nell'anno in corso questo divario rispetto all'anno precedente non si è accorciato, cosa che invece è accaduta in quasi tutti i Paesi dell'area OCSE. Siamo il Paese con il più alto tasso di abbandono scolastico. Siamo il Paese con il più basso tasso di giovani laureati. I dati di Almalaurea dello scorso anno ci dicono che oltre il 31 per cento dei laureati, a distanza di un anno dalla laurea, non ha ancora trovato un lavoro. Ora, si può affrontare il tema con dei *bonus*, si può affrontare il tema pensando di abbassare la soglia dell'elettorato attivo (tesi originale, diciamo così, ma comunque legittima); il punto di vista di Forza Italia per quanto riguarda l'occupazione giovanile

e scolastica è una necessità e questo Governo lo sta facendo. Il terzo punto è cercare di semplificare il più possibile l'accesso al mondo del lavoro per i giovani: è qui che va a battere questa norma, che è una piccola rivoluzione nel mondo del lavoro e consente di evitare una lunga attesa tra il momento della laurea e quello dell'abilitazione professionale, evitando quindi ai giovani di dover sostenere esami di stato per poter entrare poter entrare legittimamente e a testa alta, nel mercato del lavoro, superando quella fase di passaggio che spesso viene sfruttata dal mondo dell'impresa, con *stage* o altro Grazie di laurea ci sia al tempo stesso l'abilitazione professionale. Questo riguarda tante professioni, che mi piace elencare per chiarezza di chi ci ascolta: la professione di odontoiatra, di medico veterinario, di psicologo, di farmacista, di geometra, di agrotecnico, di perito agrario, di perito industriale, di chimico, di fisico e di biologo. Si tratta, colleghi, della prima riforma ordinamentale proposta dal Governo al Parlamento nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La missione 4 è un grande cambiamento. Benedetto Croce diceva che per risolvere i loro problemi i giovani devono fare solo una cosa: aspettare. Aspettare di diventare, a loro volta, adulti.

2008 le aspettative di benessere crescente sono un lontano ricordo. Sappiamo tutti (tutti quelli che hanno figli o nipoti) che tendenzialmente le condizioni di vita dei giovani oggi saranno peggiori rispetto a quelle che furono le condizioni di vita, di occupazione e di retribuzione dei loro genitori. Il tempo è forse il valore più prezioso di quest'epoca: consentire quindi ai giovani laureati di risparmiare tempo prima di accedere al mercato del lavoro è il regalo più grosso è più concreto che gli si possa fare. Non sarà questo a risolvere il tema della disoccupazione giovanile, ma sarà senz'altro questo a creare le condizioni perché quel *gap* tra noi e gli altri Paesi europei per quanto riguarda la disoccupazione giovanile progressivamente si accorci. Per questo motivo il Gruppo

la sfera dell'educazione e della formazione di uno studente o di una studentessa e il mondo del lavoro sempre più integrato ed efficace, è una scelta lavoro sempre più integrato ed efficace, è una scelta corretta e persino necessaria per un Paese che ha bisogno di compiere lo sforzo di immaginare se stesso nella stagione che si sta dispiegando davanti a noi. In fondo,

che possa avere la speranza di un futuro per sé, senza che questa passi attraverso un investimento solido, inequivoco e determinato sul capitale umano, quello che possiamo considerare l'elemento principale che può rendere un Paese diverso da un altro, proprio perché ritrova la sua vocazione dentro la divisione internazionale del lavoro. una discussione di carattere generale che abbiamo il dovere di affrontare anche in relazione alle scelte che stiamo compiendo: il capitolo - per usare un'espressione che non lo contiene, proprio per la sua dimensione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non solo. qualsiasi scelta che sta su questo terreno, almeno da parte dei senatori seduti in questa porzione dell'Emiciclo, ci sarà una grande disponibilità e soprattutto una grande curiosità,

rendere alcune classi di laurea immediatamente abilitanti all'esercizio della professione sia non solo un *escamotage* semplificativo (e di semplificazione abbiamo bisogno), ma sia qualcosa che rende più moderno e più contemporaneo il sistema della formazione universitaria e ci mette nelle condizioni di dotarci di un obiettivo ambizioso, che è quello di stringere i bulloni nel rapporto tra i percorsi di formazione, i percorsi professionalizzanti e la professione, il mondo del lavoro. Tutto ciò sapendo naturalmente che intanto le classi di laurea, quindi i corsi di studio interessati da questa riforma, dovranno inevitabilmente farsi attraversare da un processo di rivisitazione persino molto radicale: non sarà, infatti, la stessa cosa formare uno studente uno studente o una studentessa che, anziché fare l'esame abilitante dopo la laurea, fa coincidere l'ultimo dei suoi esami esattamente con il passaggio in cui viene abilitato alla professione. Pertanto, inevitabilmente, se non vogliamo fare qualcosa di il percorso di studi di quella studentessa o di quello studente dovrà essere attraversato, informato da una modifica sostanziale e questo sarà il compito del sistema universitario e naturalmente di noi legislatori che dovremo accompagnare questo processo. Tutto ciò, però, anche sapendo che non basta questo strumento di semplificazione, che io ritengo utile: non è con un'etichetta più immediata e più rapida che ci si appiccica addosso che noi mettiamo i laureandi immediatamente nelle condizioni di poter esercitare fino in fondo la propria professione. Dico ovviamente una banalità: c'è bisogno di un meccanismo di accumulazione di esperienza, ma anche di tanta passione da parte degli studenti che scelgono una professione perché è quella che vogliono fare e non come alternativa residuale

della pandemia, quando sostanzialmente abbiamo permesso che gli studenti di medicina laureati potessero svolgere immediatamente un lavoro che è stato prezioso (per usare un eufemismo), che ci ha consentito di salvare vite umane, di tirarci fuori da una condizione di grande difficoltà. Quella scelta è stata felice nel dramma; mi perdoneranno i colleghi per l'ossimoro, ma di fatto si è trattato di questo, cioè di consentire a giovani donne e uomini di mettersi immediatamente nelle condizioni di poter di poter svolgere una funzione in generale molto importante, in quel momento fondamentale per uscire dalla crisi sanitaria. Pertanto, allargare questa possibilità ad altre classi di laurea mi pare una scelta sensata, che va nella giusta direzione, che rende il nostro sistema formativo universitario più adeguato, più all'altezza, più contemporaneo. Io penso che, proprio in fase di implementazione innanzitutto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, occorra avere in mente esattamente questo obiettivo, cioè come riportiamo al centro della nostra agenda le questioni che riguardano in generale i percorsi di educazione e di formazione, la ricerca, l'innovazione, la scuola scuola al centro della dell'agenda politica; inoltre, per ciascuno di questi tasselli fondamentali occorre avviare un processo di riforme che abbia l'ambizione di riportare questo Paese nel posto che merita, cioè nel futuro. *(Applausi)*. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà. dal suo inserimento fra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che devono essere tassativamente approvati entro il 31 dicembre prossimo. Tale scadenza ha profondamente inciso sull'*iter* di questo disegno di legge, contrassegnato da un'urgenza che ha imposto scelte dettate dal senso di responsabilità. Mi riferisco alla scelta di approvare, in Commissione al Senato,

che ha determinato e determina tutt'ora la presenza del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione in questo Governo, le osservazioni del nostro Gruppo all'attuale formulazione del provvedimento in esame sono state tradotte in ordini del giorno cui il Governo auspichiamo dia prontamente seguito, così come dovranno essere emanati i provvedimenti attuativi della legge in discussione. Occorrerà, inoltre, intervenire con tutte le modifiche normative che sarà necessario apportare, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, la cui riforma non appare più procrastinabile, alla luce dell'approvazione del provvedimento oggi all'esame di questa Passando al merito del disegno di legge, è necessario ed urgente semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, facendo in modo che l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincida con l'esame di stato, perché in tal modo si riducono notevolmente i tempi per accedere al mercato del lavoro. Fino ad oggi, il percorso per accedere ad una professione dopo la laurea sembra concepito come una gara ad ostacoli, a causa delle complesse pratiche burocratiche da espletare e dei tempi troppo lunghi che un giovane deve aspettare per vedere evase le varie richieste. Questo, oltre a costituire un disincentivo per la scelta professionale, finisce a volte per limitare i giovani nella costruzione del loro futuro, nel loro consolidamento come donne e uomini in grado anche di strutturare una propria famiglia. Questo disegno di legge, ove venga attuato come auspichiamo e con i correttivi che si renderanno necessari, è un primo passo per permettere ai giovani di arrivare prima, di vedere concretamente realizzato il proprio futuro in tempi più rapidi ed offre loro la possibilità di scegliere come rapportarsi al mondo del lavoro e alla loro vita. La *ratio legis* condivisibile consiste quindi nell'arrivare, dopo anni di studi, ad un accesso più immediato, senza però tralasciare l'aspetto pratico e tecnico della formazione. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studi interessati dall'intervento normativo viene garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico ed una verifica della stessa. Per conseguire tali obiettivi, è necessario che il mondo dell'istruzione interessato da questo provvedimento diventi a tutti gli effetti il pilastro delle professioni che si andranno a svolgere, con un'accelerazione di impronta pratica che possa costituire una vera anticipazione di quella attività che i giovani si accingono ad intraprendere. Ci attendiamo, a tal fine, che si costituisca una vera ed efficace sinergia tra tutti i soggetti interessati, perché solo attraverso l'ascolto, lo scambio, la collaborazione di idee e l'esperienza di chi vive quotidianamente il mondo dell'istruzione e degli esponenti del mondo delle relative professioni si potrà realmente iniziare un percorso di cambiamento. Ai dubbi sollevati riguardo al disegno di legge in esame relativi ad una disparità di trattamento, riteniamo che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 6 costituiscano una risposta. Per quanto sopra esposto, auspichiamo che il Parlamento approvi quest'atto in via definitiva ed annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

l'istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È attraverso l'istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico o che il figlio di un minatore può diventare dirigente della miniera o ancora che il figlio di un bracciante può diventare il Presidente di una grande Nazione. Queste erano le parole pronunciate dal Presidente di una grande Nazione, Nelson Mandela. Istruzione e ricerca sono, infatti, i settori con il più alto fattore di rendimento eppure l'Italia ha ha tagliato in questi anni proprio in questi settori in cui non bisognerebbe mai smettere di investire. Ancora paghiamo cara sulla nostra pelle quella stagione di tagli tagli praticati dal Governo Berlusconi nel 2008 (che ha tagliato un miliardo di euro al fondo ordinario per gli atenei e 8 miliardi alla scuola), dai Governi Monti, Letta e Renzi. Per effetto di questi tagli l'Italia è stato l'unico Paese dell'area OCSE che per ammortizzare la fase di maggiore recessione ha tagliato proprio in università e ricerca, in controtendenza rispetto invece a tutti gli altri Paesi più lungimiranti, Germania in testa, che in quei settori hanno investito. I tagli, il blocco del ricambio generazionale, la concentrazione del sistema accademico in pochi poli, hanno fatto sì che il nostro corpo docente universitario sia ormai il più anziano d'Europa e che il 50 per cento del corpo docente delle nostre università sia costituito da personale precario.

per ogni dottore di ricerca l'Italia investe 400.000 euro e poi solo uno su tre dei nostri dottori di ricerca può lavorare in Italia. Il Parlamento, però, è impegnato da tempo a invertire questa rotta e la legge che oggi stiamo approvando ha proprio lo scopo di semplificare l'abilitazione all'esercizio delle professioni rendendo le lauree abilitanti. Come è stato ricordato dai miei colleghi che sono intervenuti, in effetti già da inizio pandemia con il decreto cura Italia abbiamo reso abilitante la laurea in medicina e chirurgia perché in quei mesi avevamo bisogno di immettere risorse nel nostro Servizio sanitario nazionale, che era a corto di personale. Oggi, dopo più di un anno dall'approvazione di quella legge, stiamo estendendo le lauree abilitanti ad altre discipline scientifiche quali, ad esempio, farmacia, chimica, tecnologie farmaceutiche, odontoiatria, medicina veterinaria, psicologia e diverse lauree tecniche in edilizia, in tecniche agrarie e forestali, tecniche industriali. Sono tutte lauree che già prevedono - questo è importante ricordarlo - un tirocinio di valore professionalizzante con un esame conclusivo del tirocinio, che da oggi costituisce anche l'esame di accesso all'esercizio della professione, proprio nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e in continuità con la missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie a questa semplificazione stiamo riducendo quel periodo che andava da sei tra la laurea e l'abilitazione e stiamo velocizzando l'accesso dei nostri giovani al mercato del lavoro. Parliamo di professionisti in aree tecniche che saranno funzionali in ambito economico, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di superbonus, di efficientamento energetico, di protezione dal rischio sismico e di sicurezza alimentare che serviranno al Servizio sanitario nazionale. Era il quarto secolo avanti Cristo quando Diogene di Sinope diceva che le fondamenta di ogni Stato sono l'istruzione dei suoi giovani e, invece, per un decennio l'Italia ha ritenuto superfluo investire in istruzione. Il Parlamento, però, ha messo l'istruzione e la ricerca finalmente al centro dell'agenda politica. In questi anni abbiamo lavorato su tre pilastri. Il primo è rafforzare il diritto allo studio: abbiamo innalzato la soglia ISEE al di sotto della quale non si pagano le tasse universitarie da 13.000 a 23.500 euro, per permettere a tutti gli studenti meritevoli di studiare all'università. Abbiamo colmato l'imbuto formativo dei giovani medici: nel 2018 avevamo solo 6.200 contratti di formazione specialistica, mentre Stiamo lavorando alla riforma del dottorato di ricerca e ringrazio di nuovo la ministra Messa, perché le borse di dottorato sono passate da 9.000 a 20.000.

Stiamo lavorando alla riforma degli istituti tecnici superiori e in legge di bilancio abbiamo previsto ingenti risorse in ambito di università e ricerca, per stabilizzare finalmente i tanti precari storici della ricerca e per permettere a tutti i giovani che scelgono questa strada di poter avere dei fondi per svolgere progetti innovativi. Tutte queste misure sono indirizzate a realizzare quella visione di futuro che il MoVimento 5 Stelle ha ben chiara. La visione di un Paese che valorizza i giovani, che permette a tutti, soprattutto a chi proviene da famiglie in condizioni economiche svantaggiate, di studiare, realizzare i propri sogni e mettere a frutto i propri talenti. Un Paese che ha consentito a me, che sono figlia di un artigiano, grazie a borse di studio, di potermi laureare in medicina e oggi di sedere qui in Senato, dove difendo proprio il diritto allo studio e al riconoscimento del merito. Un Paese, Presidente, che deve tornare a correre partendo proprio dagli investimenti in ricerca. Per tutti questi motivi, annuncio con orgoglio il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Desidero esprimere, qui nell'Aula del Senato della Repubblica, la mia e la nostra solidarietà a un giornalista che per il suo straordinario lavoro è stato ed è tutt'ora minacciato di morte dalla 'ndrangheta e dalle mafie del narcotraffico internazionale. La sua tutela è stata portata al massimo livello dalle Forze dell'ordine, ventiquattr'ore su ventiquattro. Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai 3 e direttore e conduttore di "Report" che ho conosciuto più di vent'anni fa, è sempre stato un giornalista caparbiamente determinato nella sua indagine, nella ricerca e nel raggiungimento della verità fattuale, con la massima onestà intellettuale e deontologica. Lo dimostrano - credo - i potenti e tanti nemici che oggi mettono in pericolo di vita lui e tutta la sua famiglia. Credo che possa essere di esempio per tutti e non solo per il giornalismo investigativo, così come lo sono tutti i giornalisti sotto scorta minacciati dalla mafia. Credo anche che «Report» possa essere valorizzato dall'azienda RAI

e sulla nomina di dieci nuovi direttori, che avranno un grande potere che potrà anche limitare la libertà editoriale di programmi d'informazione importantissimi come «Report». L'appello è pertanto per la massima libertà di questi giornalisti e

Giuseppe Gibboni, Alexander Gadjiev e Leonora Armellini: voglio che questi nomi risuonino in quest'Aula. A molti forse questi nomi non diranno nulla, ma il maestro Giuseppe Gibboni, a soli vent'anni, è il quarto italiano nella storia ad aver vinto la cinquantaseiesima edizione del Premio Paganini. Prima di lui, il prestigioso riconoscimento era stato attribuito agli italiani Salvatore Accardo nel 1958, Massimo Quarta nel 1991 e Giovanni Angeleri nel 1997.

Il primo, nato nel 1994 a Gorizia in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni e suona sui palchi più importanti al mondo, riscuotendo ampio successo e commenti positivi di critica. Leonora, classe 1992, dieci anni fa è stata premiata allo stesso concorso «Fryderyk Chopin» di Varsavia per la straordinaria musicalità e la bellezza del suono. Questa competizione, qualche giorno fa, l'ha vista vincere un quinto premio, che vale oro, consentendole di approdare alla finale di uno dei concorsi più importanti al mondo. Oggi voglio dedicare questo intervento di fine seduta proprio a loro, ai nostri ragazzi che portano l'arte italiana in giro per il mondo e a tutti i musicisti che con tenacia, perseveranza e abnegazione ci rendono orgogliosi di essere italiani. un solo rammarico, che è insieme anche un impegno: alla notizia dei prestigiosi premi vinti dai nostri connazionali non è stato dedicato abbastanza tempo da parte dei canali d'informazione. È un peccato non celebrare successi di tale portata

anche un impegno: che il diritto all'arte sia garantito a tutti i ragazzi e non solo ai figli dei musicisti, così come ci detta la nostra Costituzione. Questo è un impegno che dobbiamo assumere insieme in quest'Aula. *(Applausi)*.

nel carcere di Torino, che, sottoposto a turni massacranti, è al limite delle forze. Tale situazione è stata denunciata il 19 ottobre congiuntamente dalle sigle sindacali

siamo nel caos più totale. Sottolineo che già in passato abbiamo presentato diverse interrogazioni sulla disorganizzazione e sul disagio del personale di Polizia penitenziaria, che opera nel carcere di Torino. L'ultima è del 21 settembre, a firma mia e di altri colleghi, ma le segnalazioni e i comunicati ormai congiunti di tutte le sigle sindacali continuano ad arrivare giornalmente. Questo significa che le forze della Polizia penitenziaria sono arrivate allo stremo. Tensione, stanchezza e stress psicofisico, già evidenziati ad alti livelli nei mesi passati, si sono visti ulteriormente aggravati a ottobre per mancanza di personale, personale, richiami in servizio nonostante i riposi programmati e i turni cambiati o completamente stravolti senza preavviso. Addirittura, sembra che potrebbero essere a rischio le imminenti ferie del periodo natalizio. Nel carcere di Torino, quindi, il personale è allo stremo, tanto che si prospetta un incremento della pericolosità per tutti, e la salute del personale di Polizia penitenziaria femminile e maschile è a serio rischio. Il tema della riforma della giustizia è stato anteposto nelle scelte del Governo in tema di PNRR e ci è ben nota la sensibilità del ministro Cartabia sull'argomento, quindi a un pronto intervento non solo nei piani futuri, ma anche e soprattutto nell'immediato, nel carcere di Torino, ma anche in tutta Italia. È recentissima la notizia di sette agenti di Polizia penitenziaria feriti e intossicati a Como, a causa della reazione violenta e incendiaria di un detenuto; gli episodi non si contano più. Chiediamo quindi di aumentare l'organico della Polizia penitenziaria, magari già in occasione della prossima legge di bilancio.

che abbiamo depositato il 15 luglio scorso durante la seduta n. 347, avente ad oggetto l'obsolescenza degli impianti per la radioterapia oncologica. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza viene stabilita